finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

del limite degli emolumenti e delle retribuzioni per i dirigenti e per il personale della RAI.

alle retribuzioni dei vertici della RAI trovi spazio all'interno di questo provvedimento. Per la verità, la questione era già stata sollevata un po' di tempo fa in Commissione di vigilanza e, su iniziativa del Partito Democratico, la Commissione di vigilanza aveva approvato all'unanimità una risoluzione che impegnava adottare i 240.000 euro come limite massimo per la remunerazione dei vertici della RAI.

un limite analogo. Ciò non toglie che ritengo opportuno che tale limite sia stabilito sin da ora all'interno della legge di cui stiamo parlando. Per questo motivo ho presentato,

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 1.*bis*.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-*bis*.l non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

Signor Presidente, alla luce delle parole del relatore, che presenta questo nuovo emendamento, anche se sappiamo che la materia non è nuova perché ci sono altri emendamenti

parere contrario.

sulle scelte che abbiamo fatto o le diano per acquisite anche personalità di forze che queste scelte hanno contrastate o non hanno mai assunte. Non è vero che l'emissione di *bond* o di obbligazioni RAI sia la prima operazione in questo senso che fa l'azienda: la prima operazione è stata la quotazione in Borsa di RAI Way. la quotazione in Borsa di RAI Way. Al riguardo, mi piacerebbe riprendere parole che ho sentito anche in quest'Aula, con previsioni nefaste di esiti infausti e di crolli, la privatizzazione di RAI Way ha reso dinamico un soggetto pubblico in un mercato che fino a quel momento era lasciato unicamente all'attività di un noto soggetto privato ed è questa la prima operazione operazione finanziaria che ha contribuito ad intervenire sul debito e a ristrutturarlo. Mi spiace che una persona che giudico competente come il presidente Tremonti non riconosca il merito di una dirigenza come quella di Luigi Gubitosi, che ha fatto un'operazione meritoria sulle finanze e sull'aspetto gestionale della Poi ci sono le altre scelte. Noi discutiamo - e il presidente Calderoli si spingeva addirittura a ipotizzare le cifre del maggior introito - del canone,

stava lavorando in quella direzione. Personalmente, ho sempre ritenuto che il percorso corretto fosse quello quello di valorizzare il lavoro di ciascuno di noi, per il ruolo che ha, negli organismi di cui fa parte e se la Commissione parlamentare di vigilanza ha un senso, lo ha esattamente in questa direzione: nel dare indicazioni e valutare i risultati. Penso sia negativo che diamo continuamente la sensazione di un eterno nuovo inizio, come se ogni volta, su una spinta emotiva, cancellassimo noi stessi le cose che facciamo anche all'unanimità. Pur tuttavia, pienamente consapevole del segnale che si vuol dare e anche consapevole del fatto che, come il presidente Renzi ha già fatto se non vi fosse stata una risposta convincente degli organi dirigenti della RAI, il Governo era pronto a intervenire in sede di legge di stabilità, non ho alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento del relatore, che apprezzabilmente cerca di ricostruire su questo quell'unità che si era determinata nella Commissione bicamerale di vigilanza.

per la propria competenza, dal Governo, dal Parlamento, dalla maggioranza e dalle diverse gestioni della RAI (mi riferisco, in particolare, a a quella della presidente Tarantola e del direttore Gubitosi), i risultati raggiunti e le scelte che hanno portato la RAI a questo punto. Tuttavia, gli emendamenti non vanno in una direzione opposta, per cui, se i Gruppi (a cominciare, evidentemente, dal Partito Democratico e dagli altri Gruppi di maggioranza) ritengono utile un ulteriore forte segnale in questa direzione, il Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire a questo invito.

Vorrei richiamare la sua attenzione sull'intervento del rappresentante del Governo, che è andato ben oltre l'espressione del parere e, a mio giudizio, riapre, come prevede il nostro Regolamento, la possibilità

ho prospettato, applicato in questa direzione, naturalmente il nostro Gruppo si riserva un intervento sulle dichiarazioni del Governo.

Signor Presidente, sarò telegrafico e recupero le osservazioni del presidente Gasparri. Anche al fine di agevolare il lavoro del Presidente della 5ª Commissione,

ostruzionistico da parte delle forze di opposizione - ha parlato Gasparri e ora parlo io - sul tenore e il contenuto

A uno sguardo d'insieme, certamente l'emendamento è di risparmio e anche i subemendamenti mi sembra vadano tutti nella stessa direzione

Giacomelli, lei ha vantato giustamente la quotazione di Rai Way, che ha consentito alla RAI di controllare la maggioranza di Rai Way e di incassare i soldi. Lei ha di fronte colui che impedì la svendita di Rai Way

faccio il caso dell'avvocato - può avere un pagamento che le tariffe professionali fissano. Ma noi vogliamo evitare che un consulente della «Domenica Sportiva»

Per quello vale comunque il tetto stabilito per i collaboratori e i consulenti, salvo che le tariffe della professione - questo dice il subemendamento - stabiliscano i casi che ovviamente l'evidenza dei fatti regolamenterà. Ho fatto l'esempio dell'avvocato che fa vincere alla RAI una causa internazionale

Signor Presidente, farò ancora una volta un intervento telegrafico, perché mi sembra giusto fermare un po' le idee su quanto sta accadendo. Ho la sensazione - e in tal senso mi piace sottolineare il termine positivo della circostanza - che ci sia una riconciliazione, per così dire, fra quello che accade in Commissione di vigilanza RAI e quello che accade in quest'Aula,

voto. Ritengo però giusto evidenziare come la volontà delle forze di opposizione sia stata riprendere un concetto che in precedenti legislature lo stesso Partito Democratico aveva individuato ed esposto. Poi, di recente, quella tenace volontà di

la disparità di trattamento esistente tra i vari *civil servant* che si adoperano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e del sistema radiotelevisivo, sia un fatto assolutamente positivo. Mi fa piacere apprezzarlo anche come segno di uno sforzo

Forza Italia voterà a favore dell'emendamento del relatore, il quale non soltanto è stato modificato da un nostro emendamento che ha avuto parere favorevole, ma addirittura origina da emendamenti

per tutti i rami della pubblica amministrazione debba valere anche per quello più visibile che è la RAI, e debba valere per tutti quanti. matrice, frutto di una battaglia lunga, non certo iniziata con il provvedimento in esame, per uniformare e rendere trasparenti i redditi della RAI, che a lungo non lo sono stati.

a utilizzare una serie di limiti legislativi e di codicilli: così si disse, non più tardi di un paio di mesi fa.

che altrimenti avrebbero permesso di proseguire sull'incerto terreno delle interpretazioni legislative, che hanno portato non

modo di intendersi sulla sostanza delle cose e sulla bontà delle correzioni, che anche in Assemblea possono avvenire, quando ciò si rende necessario.

Voglio dire a quest'Assemblea e ai colleghi che poco fa si sono scaldati che in politica contano i fatti. E questa maggioranza parlamentare sta dimostrando con i fatti la possibilità di incidere e di cambiare le cose. L'emendamento di oggi

ha regnato in RAI una stratificazione di stipendi cresciuti a dismisura senza giustificazione e, molto spesso, assegnati

saranno in grado di condizionare tutto il mercato delle comunicazioni e di avviare un procedimento virtuoso per cancellare anche le pagine nere che prima ho citato. Per tornare a dare

che questa maggioranza parlamentare e il Partito Democratico hanno voluto con forza. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Voglio ricordare al collega Airola che, ancora prima del suo emendamento, c'erano sulla trasparenza gli emendamenti firmati dai senatori

in RAI gli stipendi inferiori ai 2.000 euro, perché bisogna dire basta anche a una RAI che è debole con i forti e forte con i deboli, come i tanti precari che la mandano avanti. apprezzo particolarmente l'emendamento del relatore Cociancich perché un punto politico lo sostiene: recepisce per intero il dispositivo della Commissione di vigilanza, che il Partito Democratico ha voluto con forza, ma che è stato votato da tutte le forze parlamentari. In questo c'è un tratto distintivo di un lavoro parlamentare che vuole essere unitario, di una iniziativa politica che vuole essere forte, ma al tempo stesso fortemente unitaria.

si sta lavorando, per avere trasparenza e tracciabilità su tutto, su tutti gli stupendi (anche quelli degli artisti), su tutte le collaborazioni (anche quelle dei produttori), per rompere vincoli monopolistici che molto spesso condizionano troppo la RAI e non permettono l'accesso

apprezzo questo dietrofront, lo apprezzo davvero molto, perché noi quel che dovevamo fare lo abbiamo fatto a suo tempo chiedendo alla Camera l'emendamento che evitava la postilla-raggiro, ossia quella che consentiva alla RAI di distribuire prebende enormi. Allora il PD votò contro, ma oggi ripara quel danno, e io ne sono contento. Pertanto mi asterrò, perché voglio lasciare al Partito Democratico tutto il merito di passare la paletta dove il Movimento 5 Stelle ha indicato di pulire.

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'informazione rappresenta - lo abbiamo visto proprio nell'ultima parte della discussione che si è tenuta in quest'Assemblea - un segmento fondamentale della vita sociale ed economica di ogni comunità. Può sembrare inutile sottolinearlo, ma voglio ricordarlo ugualmente anche a me stesso perché stiamo vivendo un momento molto delicato. Pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità sono principi cardine che hanno formato e formano ancora oggi un dibattito che, purtroppo, nell'ambito della Commissione di vigilanza RAI si è vivacizzato oltre quel perimetro di civiltà che pure dovrebbe appartenere a Commissioni che svolgono ruoli e compiti che - per la natura stessa dei principi che in quella sede si difendono le fondamenta di uno Stato democratico, soprattutto con riferimento proprio al principio dell'informazione. Quel che succede in questo periodo intorno alle vicende che interessano il servizio pubblico televisivo è emblematico di una situazione che sembra andare deteriorandosi a discapito di un'informazione plurale e corretta. Lo squilibrio, la disparità nell'ambito dei tempi e dei contenuti, per esempio, destinati al quesito referendario che forma oggetto di una modifica costituzionale di particolare rilievo per gli assetti democratici del Paese, sembra non interessare le forze di maggioranza e il Governo. Eppure si tratta proprio di incidere su quei poteri dello Stato che sono disciplinati dalla nostra Costituzione, ma che trovano un dibattito assolutamente asfittico e insufficiente a far emergere la complessità e la delicatezza dei temi in discussione. Abbiamo di conseguenza un'informazione edulcorata, non veritiera e insufficiente. È evidente che la libertà di stampa è una delle garanzie primarie di ogni Stato di diritto, poiché essa garantisce ai cittadini e a tutti i loro organi rappresentativi l'esercizio della libertà libertà di espressione, la salvaguardia della pluralità delle idee ed è l'asse portante del controllo del potere dello Stato.

dopo Paesi come il Nicaragua, l'Armenia e la Moldavia. Al di là di questa sconsolante constatazione riguardo al livello di tutela di un diritto così importante in un Paese come il nostro, tutti noi ci rendiamo conto che il settore Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare interviene quindi su uno dei temi di maggiore attualità, attualità, ma nel quale si registrano ancora numerosi punti di criticità. Per questo motivo ci saremmo dovuti trovare qui oggi a esaminare un testo in dare risposte più adeguate ai numerosi interrogativi e ai punti di criticità che abbiamo cercato di evidenziare nella discussione generale e di affrontare attraverso proposte emendative che non sono state tenute in considerazione. Abbandoniamo la dimensione anacronistica del sistema dell'informazione, che a noi sembra l'approccio con cui questo disegno di legge viene affrontato. una nota di apprezzamento nei confronti del relatore, che soprattutto su alcuni argomenti ha mostrato una particolare sensibilità, e anche allo stesso Governo che, attraverso il sottosegretario Giacomelli, ha recuperato un atteggiamento permeabile, nel concreto più incisivo, più disponibile, perché all'ascolto non ha fatto seguito l'accoglimento di almeno una parte di quegli emendamenti che probabilmente fra qualche anno, fra qualche mese addirittura, ci troveremo a dover riproporre per superare i punti rimasti irrisolti. Abbiamo cercato di intervenire con un'attività emendativa come al solito non ostruzionistica e puntuale, con tutte le difficoltà che anche il dibattito ha segnato. A questo punto mi fa piacere evidenziare quello che avviene sul *web*, uno spazio costellato da una continua ricerca di notizie da parte di utenti che spesso si affidano a fonti non sufficientemente accreditate (fonti In questo panorama si continua a ragionare in termini riduttivi e cristallizzati e, al tempo stesso, non si recupera non si recupera il senso di quella responsabilità che pure avrebbe giovato a superare qualche nodo ideologico, così come è emerso anche in alcuni interventi dei colleghi di maggioranza. Così, il grande classico è la distinzione tra la RAI e le TV locali, tra la piccola e la grande editoria. Dovremmo riuscire a considerare questo panorama in maniera univoca, organica ed armonica. Dovremmo farlo assumendoci la responsabilità del cambiamento attraverso una strategia normativa e culturale che possa costituire una svolta una svolta veramente decisiva per il settore. Invece cosa si fa? Si continua ad utilizzare lo strumento della delega al Governo, che, ancora una volta, impedisce al Parlamento di intervenire e modificare, migliorandolo, un testo che lascia molto a desiderare. Ribadiamo pertanto, da una parte - ancora una volta - la nostra ferma contrarietà all'utilizzo dello strumento della delega in modo smodato ed eccedente le effettive necessità, non solo come opposizione, ma prima di tutto come componenti di un Parlamento che deve recuperare la sua funzione primaria e il suo ruolo al servizio della nostra comunità. Dall'altra parte, riteniamo che il provvedimento in esame non sembra raggiungere l'obiettivo

Sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti - si tratta di un aspetto che mi piace evidenziare - nella parte riguardante il numero dei componenti del Consiglio, che si riduce a 60 rispetto a quello attuale di 144, e il giusto riequilibrio della rappresentanza a favore dei professionisti, siamo soddisfatti di poter dire di essere stati tra i proponenti e di aver dato, in modo motivato e puntuale, un contributo all'accordo raggiunto. Ma credo che ciò non basti. Ci sono molti buchi neri. Avremmo voluto molto di più e purtroppo non possiamo accontentarci di meno. Torno ad apprezzare il lavoro che si è fatto soprattutto in conclusione, con l'approvazione dell'emendamento sui tetti, ma credo che questo sia assolutamente insufficiente a consentirci quello che avremmo pure voluto fare e cioè esprimere un parere

fiducia perché si recuperi di più e meglio nel dibattito dell'Assemblea quell'elemento che fonda la funzione stessa dell'Assemblea, che attraverso la discussione e il dibattito tenta di individuare il prodotto legislativo migliore. Non diremo no, ma ci affidiamo all'astensione per esprimere il nostro pensiero di delusione e di auspicio che si possa fare di più e meglio per il futuro. Questo è il pensiero che esprimo a nome del Gruppo Conservatori e Riformisti.

Per questo motivo, ringrazio il sottosegretario Giacomelli e il relatore Cociancich per la collaborazione proficua e continua che hanno assicurato. Il settore dell'editoria attende da tempo una riforma organica, considerata indispensabile per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale e per invertire la tendenza negativa sul fronte dell'occupazione giornalistica. In questo senso, i dati forniti dal presidente dell'Istituto nazionale Questa riforma rappresenta un indubbio passo avanti per ridefinire le modalità del sostegno pubblico all'editoria in un'ottica di maggiore trasparenza. centrale la previsione della delega al Governo a identificare criteri e principi direttivi che colleghino l'entità del contributo alle politiche occupazionali e all'applicazione puntuale dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella fase di accesso ai contributi, la legge vuol accertare l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editoriali e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo. Si tratta di obiettivi tutti condivisibili, ma che necessitano di particolare accortezza nella loro traduzione in pratica da parte del Governo in sede di adozione dei dei decreti legislativi, tenendo conto delle nuove dinamiche socio-economiche che incidono sul settore dell'informazione e delle concrete esigenze della tutela di diritti fondamentali di professionisti che svolgono - non dimentichiamocelo mai - una funzione essenziale per la democrazia. siamo di fronte a una buona riforma, anche se alcune aspettative degli editori delle testate locali resteranno deluse. L'editore è un imprenditore e, come tale, deve necessariamente operare sulla base di attendibili piani di previsione, il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano. Se così è, la concessione del contributo non può essere un evento discrezionale e incerto. Dovrebbe essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettare le condizioni previste dalla legge. Un tempo era riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo. Poi, il fondo per l'editoria è stato progressivamente svuotato, e la mancanza di certezze ha messo in gravissime difficoltà le società editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi. La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Espressione palesemente ambigua, che non corrisponde all'esigenza, che l'editore imprenditore ha, di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione del contributo pubblico. La seconda considerazione è che il giornale cartaceo, che ha già attraversato una complessa evoluzione tecnologica,vede restringere ogni giorno le vendite e gli spazi di mercato. Anche se la sinergia con il *web* è ritenuta un valore aggiunto, forse sarebbe stato opportuno un sostegno un po' meno vincolato allo sviluppo del *web*. Dove sia la causa di questa crisi è sotto gli occhi di tutti: la congiuntura economica negativa ha infatti abbattuto il mercato pubblicitario, riducendo gli investimenti e dirottandoli, per la gran parte, verso la televisione, con ciò infliggendo un duro colpo colpo alla carta stampata, peraltro già indebolita da un verticale crollo delle vendite anche in conseguenza dell'avvento di Internet. Ci sono poi alcune criticità che abbiamo segnalato in Commissione, come la previsione che il fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della pubblicità. Si tratta, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta, e si introduce così una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva dello stesso principio di uguaglianza. Il testo uscito dalla Camera prevedeva che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, fossero escluse dai finanziamenti pubblici. Relatore e Governo - e di ciò li ringrazio - hanno accettato di prorogare di altri due anni l'accesso ai contributi per queste imprese, e questo almeno darà loro più tempo per ristrutturarsi. Purtroppo, restano escluse dai contributi le riviste scientifiche, e questo resterà un un *vulnus* per la dimensione culturale del nostro Paese. Comunque, questa riforma era necessaria e sposa, come si dice, le dinamiche della modernità. I cambiamenti intervenuti nel sistema dell'informazione hanno reso indispensabile un intervento organico che, per prima cosa, rimettesse ordine in un corpo normativo frammentato. Vanno in questa direzione i criteri premiali che incrementano le quote di rimborso per chi investe nella trasformazione digitale. Concludo dicendo che, più in generale, giudichiamo con favore la destinazione di risorse più consistenti per il settore dell'informazione la parallela attualizzazione dei criteri di assegnazione dei contributi alle imprese editoriali, in direzione di una maggiore trasparenza. Anche se l'auspicio è che il Governo, attuando la delega legislativa, dia qualche certezza in più alle imprese editrici, che hanno il sacrosanto diritto di poter sapere tempestivamente su quando e su quanti contributi poter contare. Il testo che ci apprestiamo a votare dunque è un passo in avanti per garantire il pluralismo dell'informazione. Per questa ragione, il nostro Gruppo voterà favorevolmente.

profonda e articolata, che investirà non solo la disciplina dei contributi statali ma anche temi delicati come la pensione dei giornalisti, le funzioni dell' ordine professionale e quella delle edicole. Una riforma che non terminerà con l'approvazione definitiva della legge, perché molte delle nuove norme saranno affidate a decreti attuativi emanati in seguito dal Governo. La parte più importante della riforma è, senza dubbio, l'istituzione presso il MEF del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Una volta approvata la riforma, sarà esclusivamente il Presidente del Consiglio, con un decreto, a stabilire una volta l'anno le testate che beneficeranno del contributo statale e in quale misura. Il Fondo sarà alimentato da più risorse: quelle destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, quelle per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e da una parte (con un tetto di 100 milioni di euro) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI per il triennio 2016-2018. Si è deciso poi di aggiungere anche un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, compresi quelli che operano sul *web*. l'idea di portare al Fondo il ricavato delle multe irrogate dall'AGCOM per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi. A stabilire in modo più preciso la platea dei beneficiari delle risorse saranno comunque i decreti attuativi del Governo. Condizione necessaria per il finanziamento delle imprese editrici sarà l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione come cooperative giornalistiche, come enti senza fini di lucro, limitatamente a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Nella delega, però, si prescrive che ai contributi statali non potranno più accedere gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici, le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate quotate in borsa. Restano i finanziamenti, invece, per i quotidiani e i periodici espressione delle minoranze linguistiche, per quelli destinati a non vedenti, delle associazioni dei consumatori e per i periodici italiani editi all'estero. Il contributo erogabile, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento dei ricavi della testata. La delega riduce a due anni il requisito di anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata per accedere al Fondo, oltre al rispetto del contratto collettivo di lavoro. Verranno premiate le testate edite in formato digitale dinamico e multimediale, anche in parallelo all'edizione cartacea. Sempre attraverso una delega, il Governo procederà a razionalizzare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I consiglieri saranno ridotti fino ad un massimo di 60 (due terzi professionisti e un terzo pubblicisti); un'inversione rispetto alla situazione precedente. Inoltre, sarà modificato il sistema elettorale e quello pensionistico: per i prepensionamenti ci saranno infatti nuovi requisiti La legge annuncia una ridefinizione - nella direzione di un progressivo allineamento con la normativa generale - dei requisiti di anzianità per il ricorso ad ammortizzatori sociali e a prepensionamenti per i giornalisti. Per il ricorso al prepensionamento dei giornalisti sarà previsto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri. Quanto all'esercizio della professione, la legge ribadisce il divieto assoluto per chi non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti, ma parifica le tutele per le due differenti qualifiche. Viene inoltre prorogata la durata della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. Con la riforma dell'editoria si procede ad una sostanziale liberalizzazione del sistema distributivo, con il divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne e con norme che garantiscono il pluralismo delle testate nei punti vendita, che avranno orari più flessibili e un'offerta di beni più diversificata. Dal 2017, inoltre, la parità di trattamento per le edicole, e cioè l'obbligo per i giornalai di mettere in vendita tutte le pubblicazioni che vengono mandate in edicola da grandi e piccoli editori, sarà attenuata: sarà valida infatti solo in occasione del primo lancio sul mercato delle testate. Nell'ambito della delega si prevede inoltre l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione o alle *startup* innovative. Infine vorrei ricordare come, positivamente, si prevede la riduzione a dieci anni della concessione per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ora in vigore con la RAI è di dodici anni (come previsto dalla legge Gasparri), mentre precedentemente era di vent'anni. Lo schema di convenzione, che sarà annesso alla concessione, sarà il risultato di una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. La convenzione con la società concessionaria sarà poi stipulata dal dal Ministero dello sviluppo economico.

al provvedimento, perché l'abbiamo seguito in Commissione. Ringraziamo il relatore e tutta la Commissione per lo sforzo fatto ed annunciamo il nostro voto

di domenica scorsa, versa il Centro di accoglienza richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Dal racconto del giornalista, entrato anche lui, come molti altri migranti e come i loro sfruttatori, attraverso uno dei quattro varchi aperti nel perimetro del CARA, varchi che oltretutto risulterebbero visibili dalle telecamere telecamere di videosorveglianza installate, si apprende come, oltre al sovraffollamento della struttura stessa, in essa operino indisturbati gruppi criminali che addirittura sono arrivati a spartirsi gli spazi, le abitazioni e le strutture, organizzando una sorta di cittadella in cui i migranti, in attesa di conoscere l'esito delle loro domande di asilo e di protezione internazionale, vengono indirizzati verso il lavoro nero nelle campagne del foggiano e verso la prostituzione, con metodi coercitivi violenti. Sappiamo che, dopo l'uscita del *reportage* e dopo l'appello di Eugenio Scalfari dalle colonne del quotidiano «la Repubblica», il ministro Alfano ha deciso di andare a fondo nella vicenda, predisponendo un'ispezione. Io mi chiedo, gentili colleghi, come sia stato possibile che sotto gli occhi delle Forze dell'ordine che dovrebbero sorvegliare la struttura a tutela degli stessi ospiti, degli operatori delle cooperative che lavorano presso il CARA

d'intesa contro la piaga del caporalato, imprenditori agricoli senza scrupoli attingessero a piene mani dal mercato degli schiavi, perché - scusate - non ho altro termine per definire come queste persone sarebbero state trattate dal CARA di Foggia,

luogo creato dallo Stato per accogliere e dare assistenza sanitaria, umanitaria e materiale a chi cerca un futuro migliore sul suolo italiano ed europeo. Questo è, a mio avviso, l'aspetto più terribile. Oggi ho depositato un'interrogazione in merito, sottoscritta da molti colleghi, perché non è tollerabile che in Italia non siano rispettati i diritti dell'uomo, come sancito dai trattati internazionali; non è tollerabile che in un luogo dello Stato ci siano persone in situazioni di schiavitù e sfruttamento; non è tollerabile che chi ha visto sia stato silente ed abbia lasciato che gruppi criminali agissero indisturbati; non è tollerabile che chi ha omesso di vigilare su cosa stava diventando il CARA non ne debba rispondere; non è tollerabile che situazioni come quelle del CARA di Foggia buttino cattiva luce sull'intero sistema di accoglienza del nostro Paese. Signor Presidente, ci sono stati in questi giorni dei casi di cronaca molto tristi, tragici, relativi in qualche modo ad attività di divulgazione mezzi informatici. Sto pensando al caso della giovane donna di Napoli che si è tolta la vita a seguito di un video che girava in rete o a quello della giovane ragazzina

della legge sul cyberbullismo e spinge a svolgere anche qualche precisazione perché il primo caso, quello della giovane donna di Napoli, non è certamente rapportabile al cyberbullismo nella sua reale essenza. Vi è un problema tragico e gravissimo ma si tratta di persone maggiorenni. Siccome alla Camera si sta discutendo di modificare il testo che il Senato aveva approvato sul cyberbullismo, cercando di mettere insieme un po' troppe cose che insieme non stanno, tengo a ricordare che per tutti gli studi il cyberbullismo è un che riguarda l'età evolutiva, che riguarda i minori e per il quale è fondamentale la dimensione educativa. Di conseguenza è poco opportuno, perché poco efficace, mettere insieme cose che insieme non stanno. L'auspicio è che la Camera termini quanto prima l'esame del disegno di legge, che non ne stravolga l'impostazione iniziale che questa Assemblea gli aveva dato e che si riferisce, per l'appunto, a fenomeni limitati ai minori. Purtroppo è iniziato un nuovo anno scolastico senza che questa legge abbia ancora visto la luce. Speriamo proprio che il prossimo anno scolastico

*(CoR)*. Signor Presidente, vorrei stigmatizzare una situazione che credo non debba passare sotto silenzio. Volevo sapere se la Presidenza può chiedere al Ministro degli affari esteri di venire a riferire in Aula

non immagino che siamo ritornati al periodo del colonialismo. Io credo che la nostra sia una Repubblica con una propria autonomia e che quindi vada stigmatizzato quanto accaduto proprio per instaurare dei corretti rapporti diplomatici ed evitare che nel prossimo futuro ci possano essere uscite di questo tipo che non